la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino a venerdì 8 luglio. Fermi restando gli argomenti della corrente settimana, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che l'esame delle mozioni sui flussi migratori dal Nord Africa venga posto all'ordine del giorno subito dopo le ratifiche degli accordi internazionali definite dalla Commissione esteri. Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 giugno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali risponderà ad interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, su iniziative per favorire l'occupazione femminile, sullo stanziamento di risorse per le politiche sociali e familiari e sulla gestione finanziaria degli enti previdenziali privati. La diretta televisiva avrà la durata di un'ora e trenta minuti. La prossima settimana, a partire da mercoledì 6 luglio, l'Assemblea esaminerà il decreto-legge "Sviluppo", già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Il calendario prevede sedute con votazioni fino a venerdì 8 luglio. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 6 luglio, a partire dalle ore 9,30, si procederà alla votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Questore. Una volta esaurita la chiama a inizio seduta, l'urna resterà aperta fino ad un orario antecedente la chiusura della seduta antimeridiana per dare modo a tutti i senatori di partecipare alla votazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2243 è soltanto l'ultimo dei numerosi interventi di semplificazione che si sono succeduti nella legislazione a partire dalla legge n. 59 del 1997. Frutto di uno stralcio da un più ampio provvedimento, esso è stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno del 2010. Il disegno di legge, dopo l'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento, ha quindi iniziato il suo *iter* in Senato presso la Commissione affari costituzionali il successivo 23 giugno ed è collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2010, con tutti gli effetti procedurali che ne conseguono. In Commissione, dopo la relazione del senatore Pastore, si è svolto un ciclo di audizioni informali, in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Sono stati ascoltati il Garante per la protezione dei dati personali, nonché i rappresentanti del Formez PA, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di DigitPA, della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), nonché del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali. Nell'ottobre del 2010, anche in considerazione dell'ampiezza della materia e della vastità e molteplicità dei settori su cui, nell'interesse dei cittadini, era sembrato opportuno procedere alle necessarie semplificazioni amministrative, è stato presentato un significativo *corpus* di emendamenti, sia da parte di senatori dei Gruppi di maggioranza che da parte di senatori dei Gruppi di opposizione. Nella seduta della Commissione affari costituzionali del 7 giugno scorso il sottosegretario Augello, a nome del Governo, ha presentato due proposte di stralcio dirette a ricondurre ad appositi e autonomi disegni di legge, da un lato, gli articoli da 1 a 40 e l'articolo 44 e, dall'altro, gli articoli 41 e 42. La prima proposta è stata motivata dalla circostanza che molte disposizioni del disegno di legge n. 2243 sono state inserite nel decreto-legge n. 70 del 2011, approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato e che, come Presidente, ci ha comunicato poco fa, la prossima settimana sarà sottoposto all'attenzione dell'Assemblea del Senato. Altre disposizioni, probabilmente, risulteranno sostanzialmente assorbite proprio con gli emendamenti approvati in sede di conversione in legge. La seconda proposta, invece, è volta a ricondurre a un disegno di legge specifico la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, che ha una sua specifica autonomia. In ragione della natura eminentemente procedurale della proposta avanzata dal Governo, che investe l'intero testo, dal momento che la Commissione affari costituzionali, in quella stessa seduta del 7 giugno, ha approvato le suddette proposte, ho deciso di assumere la funzione di relatore per questa specifica parte del provvedimento. Il senatore Pastore, come ha già ottimamente fatto, continuerà a svolgere tale funzione per l'esame successivo dei disegni di legge che risultino dalle deliberazioni di stralcio che l'Assemblea vorrà adottare. In proposito, desidero assicurare sin d'ora che l'esame in Commissione si svolgerà tempestivamente: in un caso senza alcun condizionamento (Carta dei doveri, articoli 41 e 42); nell'altro, non appena sarà stato convertito in legge il decreto-legge n. 70 e sarà possibile, pertanto, valutarne le interferenze con le disposizioni degli articoli da 1 a 40 nonché dell'articolo 44 e con gli emendamenti aggiuntivi. Qualora fossero approvate le proposte di stralcio, l'Assemblea potrà procedere all'approvazione immediata e distinta dell'articolo 43, che reca una delega al Governo per adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi volti a riunire in un unico codice tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione. In particolare, nel codice potranno confluire le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Nell'esercizio della delega, il Governo assicurerà il coordinamento formale delle disposizioni, risolvendo eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata in proposito. Il decreto legislativo sarà da emanare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione. L'approvazione della delega consentirà in sostanza di procedere nell'importante opera di codificazione che è stata avviata negli ultimi dieci anni e che, ormai su molte materie, si è conclusa positivamente, giungendo a risultati notevoli per qualità e rigore. Ricordo il codice dei contratti pubblici, il codice dei beni culturali, il codice del turismo, il codice dell'amministrazione digitale, il codice dell'ordinamento militare, il codice del consumo, il codice della *privacy*, il codice delle pari opportunità. Nel 2010, infine, è giunta a compimento l'importantissima opera di codificazione delle leggi sul processo amministrativo. Adesso, se il Parlamento approverà questa ulteriore delega, i cittadini e gli operatori del diritto potranno avere a disposizione, raccolta in un solo *corpus* normativo, tutta la legislazione vigente che riguarda la pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i privati, al procedimento amministrativo e alla materia del pubblico impiego.

perché il relatore ha voluto fare una relazione complessiva, ma noi dovremmo procedere anche presupponendo che l'Aula bocci lo stralcio e - quindi - la discussione generale dovrebbe avere ad oggetto l'intero

del citato codice di protezione dei dati personali, così determinando un ampliamento nell'ambito di operatività della citata disposizione, consentendo il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale, non solo mediante l'impiego del telefono, ma anche attraverso l'utilizzazione della posta cartacea. tenere conto del fatto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del diritto alla vita privata. considerare che la suddetta direttiva è volta a tutelare gli abbonati a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico - siano esse persone fisiche o giuridiche - con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, al loro diritto alla vita privata e alla riservatezza. La direttiva, inoltre, prevede che «Qualsiasi ulteriore trattamento di dati che il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base a informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica». su questo registro delle opposizioni, che è stato istituito in virtù di una legge, ci sono molte, moltissime critiche, anche da parte del Garante per la *privacy*, che le ha espresse nei giorni scorsi. Voglio anche ricordare che molti cittadini sono molestati, all'ora di cena o di pranzo, da soggetti che vogliono vendere prodotti o servizi. Il Garante per la *privacy*, rispetto al *telemarketing*, ha mosso una durissima critica nei confronti del registro delle opposizioni che, a quattro mesi dal suo debutto, sta manifestando le sue debolezze, facendo emergere limiti e difetti maggiori di quanto previsto. La settimana scorsa, nel rapporto annuale presentato al Parlamento, il Garante ha definito il *marketing* telefonico una forma inaccettabile d'invasione della propria vita privata. Il registro, che doveva essere un'innovazione legislativa, non ha incontrato il favore di chi deve vigilare sulla riservatezza dei dati personali, quindi del Garante della *privacy*. Il sistema non è la soluzione giusta per aziende e consumatori, visto il gran numero di proteste ricevute dal Garante in merito: da febbraio, sono state ricevute centinaia di proteste, più del doppio di tutto il 2010, e più del 90 per cento di tali proteste riguarda proprio la violazione del registro delle opposizioni. Molti utenti iscritti al registro continuano a ricevere telefonate promozionali. Tra i motivi del fallimento di questo registro delle opposizioni vi è la mancata definizione di responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più soggetti, dalle imprese interessate ai *call* *center*. A creare rilevanti danni all'attività lavorativa di professionisti e imprese ci sono poi gli invii illeciti di fax promozionali. Su questo fronte, il Garante ha preso, nel corso del 2010 e nei primi mesi del 2011, numerosi provvedimenti sanzionatori; presto arriveranno sanzioni pesanti rispetto al *telemarketing* effettuato in violazione della nuova normativa. Il Garante lancia dunque un monito contro la possibilità di estendere il registro delle opposizioni anche al *marketing* postale, perché questo è un Paese in cui tutti tengono famiglia e, quindi, tutti assecondanoi *desiderata* dei grandi potentati, di quelli che hanno un interesse economico. E i diritti alla riservatezza, i diritti della persona, i diritti dei cittadini, i diritti della famiglia (che non vuole essere molestata quando, durante la cena, riceve telefonate per le quali non ha mai dato autorizzazione a subire molestie telefoniche) passano sempre in secondo piano. Lo abbiamo ricordato anche in quest'Aula, quando venne approvata questa vera e propria forzatura giuridica.

su alcune questioni sollevate in merito alle carte di credito dell'American Express. Anche su questo punto, la Suprema corte dice che è inviolabile il diritto alla riservatezza, il diritto a non essere molestati con vendite nella propria abitazione a tutte le ore del giorno e della notte. signor Presidente, concludo auspicando che venga accolto questo nostro ordine del giorno del giorno G102, che impegna il Governo a voler prevedere - anche in collaborazione con gli operatori del settore e le associazioni di utenti e di consumatori - idonee modalità di garanzia e di rispetto della vita privata, della riservatezza dei fruitori dei servizi, in conformità con quanto disposto dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002. L'ordine di rafforzare l'apparato sanzionatorio per la violazione evidente dei diritti degli utenti. Concludo, signor Presidente, informando anche che vi sono alcuni siti, (ho anche prodotto alcune interrogazioni parlamentari e denunce

che sono pur evidenti, ma non possono essere preponderanti rispetto al diritto dei cittadini a non essere molestati. Signor Presidente, come sempre l'interpretazione della Presidenza è legge in questa Aula. Quindi, io mi adeguo ma, come diceva quel tale, non capisco. Non capisco perché il collega Lannutti, piuttosto che altri, siano invitati a un dibattito generale su tutto il disegno

e l'opportunità politica dello stralcio, come la sua correttezza, compatibilmente con l'insieme degli altri provvedimenti, e poi il merito dell'articolo 43, che sarà l'unico che residua alla nostra attenzione e su cui il Senato sarà effettivamente chiamato a pronunciarsi. Vero è che il Senato, la nostra Assemblea, potrebbe anche respingere la proposta della Commissione e del relatore; ricordo che è una proposta fatta propria dalla 1a Commissione, con il voto contrario delle opposizioni, su richiesta del Governo: nello specifico, del sottosegretario Augello, che era presente a nome del Governo e che ha chiesto lo stralcio. Ma in questo caso, noi avremmo dovuto comunque, a mio modestissimo avviso, discutere lo stralcio come una specie di questione pregiudiziale.

mi esprimo sulla relazione del relatore e non su un provvedimento che, su richiesta del Governo, non dovrebbe essere più alla nostra attenzione. Infatti,

Comunque sia, è stato esaminato, sono state svolte le audizioni e depositati gli emendamenti; quando però stavamo per iniziare le votazioni, il Governo ci ha chiesto lo stralcio di cui stiamo parlando. Esattamente di cosa si tratta?

si riprendono moltissime di queste norme. Addirittura il relatore, se non ho capito male, afferma

come senatori dovremmo davvero opporci a questa scelta. Praticamente andiamo a operare

con gli emendamenti che passeranno. Se salterà fuori ancora qualche articolo che proprio non sapremo dove inserire, allora la Commissione affari costituzionali del Senato farà un provvedimento *ad hoc*. Poiché le finalità del provvedimento originale erano volte alla semplificazione per le imprese ed i cittadini ed alla trasparenza delle procedure, mi chiedo se c'è coerenza tra gli obiettivi che vogliamo perseguire come Governo e come legislatori nel momento in cui abbiamo presentato questo disegno di legge e le scelte che stiamo operando con lo stralcio e le votazioni sparse in provvedimenti diversi degli articoli che invece avevano una loro organicità di obiettivo e di impostazione. Mi chiedo se c'è coerenza e e trasparenza offrendo ai cittadini norme semplificate, o viceversa sparpagliare le stesse in contenitori che parlano di tutt'altro e che renderanno oscuri i processi legislativi che stiamo per

Siamo di fronte a un caso che forse può diventare di scuola come esempio del modo di legiferare di questa legislatura.

La Commissione affari costituzionali ne ha concluso l'esame il 7 giugno 2011. Poi, nell'ultima seduta, il Governo ha presentato due proposte di stralcio:

approvato dalla Camera ed ora assegnato al Senato. La seconda proposta di stralcio è volta a ricondurre ad un provvedimento specifico la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

Ciò rende più che giustificate le proteste della collega Adamo che si chiede di cosa discuteremo, se dell'articolo 43 residuo o del problema dello stralcio.

Quindi, quella che sembra una bella semplificazione in realtà è già l'inizio di una nuova complicazione, perché bisogna ricreare tutto un cammino.

In caso contrario, evitando la soppressione, dopo che ci sarà l'approvazione con modifiche del decreto-legge n. 70 del 2011, per tutte le disposizioni doppie dei collegati stralcio si porrà la necessità di una riformulazione con riferimento al testo della legge di conversione del decreto-legge, che sarà ancora suscettibile di modificazioni fino al termine finale del 13 luglio 2011. Non solo. Non solo. Il Governo alla Camera ha blindato con la fiducia il decreto-legge n. 70 del 2011, e non è improbabile che ciò avvenga anche al Senato, data la ristrettezza dei tempi. insieme lo stralcio di 43 articoli su 44 e la loro riconsegna a un procedimento che rischia di essere barocco con la blindatura del decreto-legge n. assistiamo ad una inequivocabile e potente compressione oltre misura delle possibilità di intervento sugli argomenti in merito. Ci si dibatterà tra la costruzione di nuovi provvedimenti, la fiducia e la mancanza di tempo.

Grazie Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a discutere il disegno di legge n. 2243 in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, che arriva in Aula dopo l'esame in Commissione di merito, concluso lo scorso 7 giugno con l'accoglimento favorevole di due proposte di stralcio formulate dal Governo, di natura eminentemente procedurale. L'esigenza di accelerare l'approvazione di norme importanti per il rilancio economico, nonché l'ampiezza e l'eterogeneità della natura del provvedimento, hanno indotto il Governo a dare priorità ad alcune di esse rispetto ad altre e, riconducendole in disegni di legge autonomi, a procedere con *iter* separati. Ricordo che il provvedimento all'esame ha avuto un *iter* molto articolato e complesso, iniziato il 16 marzo 2010 alla Camera, in sede referente in prima Commissione, e concluso il 9 giugno 2010 con un testo licenziato dall'Assemblea, modificato rispetto a quello presentato, dopo un rinvio in Commissione. A circa un anno dall'approvazione da parte dell'Aula della Camera, il provvedimento arriva all'esame dell'Aula del Senato, dopo una lunga sospensione dei lavori in Commissione. Nel frattempo, l'obiettivo del Governo di uscire dall'attuale crisi e di rilanciare la crescita economica è diventato una priorità indifferibile e in particolare quello della Lega Nord di contribuire in maniera decisiva a strutturare un'efficace politica di semplificazione e regolazione dei procedimenti amministrativi e delle normative è diventato un elemento strategico non più procrastinabile. In questo contesto e in risposta a tale esigenza il Governo si è adoperato attraverso l'emanazione del decreto-legge n. 70 cosiddetto decreto sviluppo, già approvato dalla Camera dei deputati e prossimo all'esame del Senato. È ormai opinione diffusa che le lungaggini burocratiche, oltre a mortificare l'iniziativa privata, rappresentano per le imprese un onere che grava sui bilanci delle aziende in misura non inferiore

hanno un'incidenza sui bilanci delle imprese pari ad almeno il 24 per cento. Pertanto, liberare il sistema produttivo, ed in particolare quello della piccola e media impresa (settore strategico del nostro tessuto industriale, oggi purtroppo più esposto e colpito dall'attuale crisi), svincolarlo da un complesso di gravose procedure amministrative, vuol dire liberare risorse utili per il rilancio economico del Paese e per attrarre investimenti internazionali. In questa direzione, noi della Lega Nord ci siamo adoperati affinché molte norme del disegno di legge n. 2243 volte a promuovere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale, unitamente a quelle finalizzate alla realizzazione di una maggiore semplificazione delle attività economiche e sociali, con particolare riguardo a quelle riconducibili all'iniziativa privata, confluissero nel «decreto sviluppo». Esse risultano quindi già vigenti ed è molto probabile che altre verranno approvate in sede di conversione in legge. Conseguentemente a ciò si inserisce la proposta del Governo di stralciare gli articoli dall'1 al 40 e il 44 e di rimandare la valutazione di eventuali interferenze con gli stessi in seguito all'approvazione in legge del «decreto sviluppo». Ciò detto, la seconda proposta del Governo riguarda lo stralcio degli articoli 41 e 42, con i quali si conferisce allo stesso la delega per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, la quale dovrà definire i doveri generali delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini. L'intento del legislatore è quello di realizzare uno strumento normativo che definisca in maniera sistematica i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del quale lo Stato è considerato come strumento al servizio del cittadino e delle imprese ed il cittadino come utente e unico riferimento per valutare la qualità del servizio offerto. Una rivoluzione che supera l'attuale realtà di una pubblica amministrazione autoreferenziale, lenta e lontana dalla società civile, per porsi come strumento al servizio del cittadino-utente sulla base di un rapporto di collaborazione che prevede il minor aggravio possibile di oneri, adempimenti e obblighi a carico dei cittadini. Noi della Lega Nord siamo convinti che senza riforma seria della pubblica amministrazione non è possibile costruire un federalismo virtuoso basato sui principi di responsabilità e di efficienza a tutti i livelli di governo e se è vero che la bassa crescita, la competitività e la credibilità a livello internazionale del nostro Paese sono in parte anche imputabili alle inefficienze della pubblica amministrazione, allora appare ancora più evidente quanto sia importante intervenire in maniera decisiva in questa direzione. Infine, l'unico articolo rispetto al quale l'Assemblea sarebbe chiamata ad esprimersi anche nel merito, qualora venissero approvate le due proposte di stralcio formulate dal Governo, è l'articolo 43. Con esso viene data priorità e quindi immediatezza alla realizzazione di codici o testi unici finalizzati all'armonizzazione, semplificazione e snellimento di una serie di norme esistenti in materia di documentazione amministrativa. La norma infatti, cosi come riformulata dal Governo, conferirebbe allo stesso la delega di adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi per l'elaborazione di codici o testi unici di disposizioni vigenti, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi. La codificazione completa l'azione riformatrice di questo Governo iniziata con la legge n. 15 del 2009 e con il decreto legislativo n. 150 dello stesso anno, restituendo organicità, armonizzazione, coerenza e quindi facilità di conoscenza e di applicazione ad una serie di norme che si sono succedute e sovrapposte negli anni in tema di documentazione amministrativa e pubblica amministrazione. In conclusione, signor Presidente, in considerazione della rilevanza delle questioni coinvolte e della necessità di tempestività, auspico che in questa Assemblea si possa riscontrare una maggiore convergenza di quella registrata in Commissione.

Presidente, colleghi, credo che mai come in questo caso si possa dire che la montagna del lavoro di tante persone dei due rami del Parlamento, funzionari, uffici legislativi, parlamentari che si sono documentati e che hanno creduto di dover discutere un'impegnativa proposta del Governo, ha partorito un ridicolo topolino, sempre che ovviamente questa Assemblea accetti la proposta di stralcio di 43 articoli su 44 che il Governo ha chiesto di fare e che la maggioranza ha già accettato in Commissione. A questo proposito, vorrei manifestare una solidarietà personale al sottosegretario Andrea Augello, nostro collega senatore. Vede, Sottosegretario: il ministro Calderoli Grazie

lei qui, al Senato, tra i suoi colleghi, a dirci mestamente: tutto quello che avete fatto è stato inutile perché del glorioso disegno di legge di semplificazione che ha impegnato il Parlamento un anno e quattro mesi rimane un unico articolo. Che cos'è questo articolo? È una banalissima delega al Governo per scrivere testi unici compilativi e non innovativi in materie anche recentemente esaminate e trattate dal Parlamento. In base all'articolo superstite ci sono, da riorganizzare e da riscrivere, addirittura delle disposizioni che riguardano il decreto legislativo 27 ottobre 2009, cioè norme che risalgono ad un anno e mezzo fa. Allora, credo che, più che parlare di questo merito (un brutto merito e una brutta pagina di dissipazione di energie), occorra fare un riferimento a quello che ci viene chiesto circa i cosiddetti costi della politica. Chi è che paga nell'opinione pubblica il costo di un anno e mezzo di lavoro del Parlamento, parlamentari, delle Commissioni, dell'Aula, dei funzionari, degli uffici legislativi, di stampe di documenti, di audizioni, di elaborazioni concertate dei vari Ministeri? Chi è che paga questo costo della politica che oggi, con un tratto di penna e di volontà del Governo e della maggioranza, del Parlamento, sottosegretario Augello, chi lo paga? Lei, insieme al ministro Calderoli, la scorsa sessione di lavori ha stralciato una disposizione dal disegno di legge anticorruzione. Forse non era il luogo giusto ove collocarla, ma era una norma che parlava di «fallimento politico». I presidenti delle Regioni che mandavano in rosso

Da cosa conseguiva questo fallimento? Dall'aver dissipato la ricchezza del Paese in un momento in cui il Paese non può permettersi di dissipare nemmeno un euro della sua ricchezza pubblica. Benissimo, interrogatevi dopo aver votato, come voterete, lo stralcio di 43 articoli su 44, sul vostro fallimento politico.

come ha ricordato anche il collega Pardi, seppur ironicamente, dobbiamo rammentare che ciascuna delle parti che risulta da questi stralci manterrà la sua natura di provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Ovviamente il Governo non intende tralasciare in alcun modo l'*iter* di approvazione di ciascuna di queste partizioni, perché ritiene che abbiano tutte la stessa importanza. Il problema dello stralcio nasce casomai dalla volontà di far prima, e comunque, per rassicurare i colleghi (che non ne hanno bisogno, perché lo sanno benissimo), ricordo che siamo in una situazione in cui nove articoli di questo provvedimento, quindi circa un quinto dell'intera legge, com'è stato ricordato, si trovano nel decreto-legge n. 70 del 2011. Quindi, la ragione per cui si arriva a questo stralcio è che alcune parti di questo disegno di legge necessitano di una serie di deleghe, date e da dare, al Governo e, perché nell'ambito della legislatura si riesca ad arrivare in fondo a questo percorso, questa è la strada più breve, come sa chiunque conosca i Regolamenti parlamentari. Detto questo, resta anche il problema che è stato segnalato già dai tempi in cui abbiamo affrontato questo provvedimento al Senato, però di questo il Governo ha modeste responsabilità, nel senso che

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esaminati gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1 (testo 2) (limitatamente al comma 3), 6.3, 7.0.1, 8.7 (limitatamente al comma l-*ter*), 8.100 (testo corretto), 8.0.3, 9.3 (testo corretto) (limitatamente alla lettera 11.0.100 (testo 2), 19.1, 19.0.2 (limitatamente al comma 4), 19.0.4, 29.1, 40.0.300, 40.0.302 43.100/8. Esprime parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri, sugli emendamenti 2.2 (testo corretto), 2.2 (testo corretto)/1, 19.0.3 e 21.2. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.1, 7.0.2, 19.9/2 (testo 2), 31.0.1 (testo corretto) e 34.0.2 (testo corretto)/1 (limitatamente al comma 19). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 37.0.1 (testo corretto), 39.1,

42.11, 42.12 e 42.15, sui quali il parere è sospeso».

credo che l'obiezione del relatore sia dirimente da questo punto di vista. Infatti, dalla percezione evidente dei testi degli ordini del giorno, mi sembra chiaro che, qualora venisse accolta la proposta di stralcio,

risulteranno preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 40 nonché all'articolo 44.

in particolare, la presenza nel "decreto-legge sviluppo" di molte delle norme contenute nel disegno di legge di semplificazione sostanziale e i molti emendamenti approvati e che fanno parte del testo che il Senato è chiamato ad esaminare, approfondire e votare. Vorrei però ricordare ai colleghi che, al di là della particolare procedura, che non ho alcun timore a definire originale, vi è questa necessità di fondo, e soprattutto

che nell'articolo 43, salvato dagli stralci e quindi possibile oggetto di una definitiva approvazione in Aula, quanto meno per questo ramo del Parlamento, vi è una continuità nella politica di questo Parlamento e dei Governi che si sono succeduti, che va dal 1997, I Governo Prodi, fino ad oggi, IV Governo Berlusconi, e che ha attraversato vicende politiche svariate nonché situazioni normative diverse tra di loro. Si è passati dai disegni annuali di semplificazione ai testi unici misti, ai regolamenti di delegificazione, alle codificazioni, ma con il solo obiettivo di creare corpi di diritto omogenei e compatti

della giustizia amministrativa, iniziativa positivamente accolta non solo negli ambienti degli addetti ai lavori ma anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dai cittadini, dagli operatori economici

cioè di diritto sostanziale, dell'attività della pubblica amministrazione raccogliendo in un unico corpo tutte le norme le norme che interessano l'attività dei pubblici poteri che fanno capo alla pubblica amministrazione. Dunque, vi sono le leggi fondamentali inerenti alla documentazione amministrativa, anche in forma digitale (quindi il codice dell'amministrazione digitale), le norme sull'organizzazione amministrativa (quindi, l'individuazione dei soggetti che hanno le responsabilità e i ruoli per esercitare i poteri amministrativi) ed infine

che ha subito continui miglioramenti e che oggi è una legge assolutamente soddisfacente. Se un ordinamento moderno potesse disporre di un unico testo

un vantaggio sia in termini di utilità che di chiarezza per i rapporti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e per l'esercizio da parte della pubblica amministrazione

illustrerò un emendamento da me presentato a questo articolo che, proprio nell'ottica della codificazione, tende a potenziare lo strumento che va sotto il nome di "taglia-leggi" (che - molti colleghi presenti sono più consapevoli di altri - è uno strumento complesso), proprio nell'ottica di un riordino complessivo del nostro ordinamento. Se arrivassimo a produrre un codice di diritto amministrativo avremmo reso un servizio al Paese e avremmo dimostrato che questo Parlamento e la classe politica sono attenti alle vicende che si verificano nel contesto nazionale e vogliono aggiornare gli strumenti che tutti noi siamo chiamati ad applicare quando svolgiamo le nostre attività. Non è quindi un punto secondario, anche se si tratta solo di un articolo, ma

Signor Presidente, non sono sufficientemente magnanima per esimere l'Assemblea dal sentire la frase

svolto dal collega Sanna, con la sua metafora della montagna che ha partorito il topolino, abbiamo abbondantemente spiegato le motivazioni della nostra contrarietà

di un disegno di legge che introduce diverse norme sulla semplificazione che ci vedevano in parte d'accordo e in parte contrari, e sulle quali stavamo svolgendo, come è giusto, la nostra opera di proposta emendativa,

Non si sa. O dovremo fare due disegni di legge diversi in Commissione? Ciò è demandato a un lavoro

si appresta a prendere atto e a stralciare. Si vedrà che cosa succede alla fine di tutto questo percorso, e solo allora,

avevamo anche una possibilità di accordo tra maggioranza e opposizione su molte questioni. Non è il tempo che è mancato: è mancata la volontà del Governo di rispettare l'autonomia del Parlamento; e forse sono mancate anche delle idee da mettere nel "decreto sviluppo". Ci si sarà allora chiesti: cosa possiamo metterci in questo "decreto sviluppo"? ricicciare per le imprese italiane un po' di norme della semplificazione, che vanno sempre bene. Per questa ragione, il nostro Gruppo voterà contro lo stralcio.

Abbiamo ascoltato con crescente incredulità, ma anche con un certo divertimento, l'orazione del collega Pastore, il quale ci ha spiegato che, avendo "stecchito" 43 articoli, l'unico articolo rimasto è di grandissimo rilievo. Non avevamo pensato a questo aspetto, e francamente accogliamo questa sorta di suggerimento alla relatività. Ce n'è uno solo di articolo, per cui: viva l'articolo sopravvissuto! Abbiamo lavorato per mesi, anzi per più di un anno, per arrivare a una soluzione, ed ora abbiamo un articolo. Di questo parlerò in occasione della votazione

a 40, nonché all'articolo 44 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo: «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese» Il disegno di legge sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 40 all'articolo 44.

mi rimetto all'Assemblea, apparendomi un ordine del giorno assolutamente ragionevole, che il Governo potrebbe accogliere. e G102, che si riferiscono specificamente a due articoli che sono stati stralciati, invito i proponenti a ritirarli, così da discuterne nella sede opportuna, giacché qui non ce ne

di un ordine del giorno importante, come ho motivato, che riguarda la *privacy* delle famiglie e di persone che, dopo una giornata di lavoro, arrivano a casa e sono molestate al telefono da chi vuole vendere un prodotto o un servizio. Io sono disponibile anche a riconsiderare qualcosa, ma non a ritirarlo.

giorno effettivamente riferiti all'articolo e quelli di materia più generale. Comunque, dato il suo contenuto, non abbiamo problemi ad accogliere

Onorevoli colleghi, prima di porre in votazione la proposta di stralcio S41.100, presentata dalla Commissione, avverto che per effetto della sua eventuale approvazione risulteranno preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 41 e 42.

e di quello che il Governo ci ha proposto nei mesi passati e che questa maggioranza non è stata in grado di portare avanti. Ma io direi soprattutto il Governo: com'è stato già detto, noi avevamo qui in Senato, dallo scorso anno, un testo pervenuto dalla Camera

Tutte queste norme, che riguardano le imprese, i cittadini, la trasparenza (perfino alcune norme importanti relative alla salute dei cittadini) sono sono state assolutamente derubricate. Adesso, con un pasticcio alquanto confusionario, alcune di queste norme vengono introdotte nel decreto sviluppo, altre verranno messe in un altro provvedimento e altre ancora

anche la persona più semplice, ma dotata di buonsenso, a chiamare tutto ciò semplificazione. Avevate i numeri e i tempi,

Signor Presidente, ovviamente anche il nostro Gruppo voterà contro questa seconda proposta di stralcio, sottolineando il fatto che passare dalla votazione di un articolo alla costruzione di una delega al Governo per affrontare i problemi che venivano affrontati in quell'articolo, francamente, è molto difficile considerarla una semplificazione.

una delega, si ingrandisce l'idea della delega. Si va avanti con le deleghe al Governo. In questa maniera, oltretutto, il Parlamento rivela sempre

o si dà la delega al Governo per attuare delle misure che il Parlamento potrebbe approvare benissimo. Mutuando da un antico classico, questo potrebbe essere un caso di servitù volontaria delle Assemblee elettive nei confronti del potere esecutivo.

colleghi, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S41.100, le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 andranno a costituire un disegno di legge autonomo dal titolo «Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche» (A.S. 2243-*ter*). Il disegno di legge sarà deferito alle competenti Commissioni parlamentari. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 41 e 42.

di provvedere all'abrogazione di disposizioni legislative e regolamentari statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se riconducibili a disposizioni di cui al comma 17. Che cosa dice il comma 17

sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura civile, sul codice di procedura penale, sul codice della navigazione e su ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione "codice". Ove approvato, quindi, questo emendamento consentirebbe d'intervenire, attraverso lo strumento di semplificazione

Il rilievo è ancora più

in tema di semplificazione anche con regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988.

transigere, signor Presidente, e la prego di assumere una decisione chiara, espressa e motivata, stante la gravità del rilievo che ho appena formulato. il collega Legnini ha svolto alcune considerazioni, però non ha detto la cosa più importante, l'articolo 14-*quater* che viene novellato da questo emendamento si riferisce ai decreti legislativi ricognitivi di abrogazioni già avvenute (non in modo espresso, ma, come è noto, nel nostro sistema è prevista anche l'abrogazione tacita). Quindi, è uno strumento per dare indicazioni di certezza a chi si trova di fronte a leggi nelle quali siano presenti norme vive ma in realtà morte, perché abrogate implicitamente da altre norme; quindi, esso fa parte di questo filone di pulizia dell'archivio legislativo che ha portato, tra l'altro, a risultati estremamente positivi. Infatti, la procedura sulla quale interviene questo emendamento, ampliando i termini della delega e consentendo al Governo un lavoro anche più approfondito e più diffuso, ha portato finalmente il nostro sistema istituzionale a conoscere la cosa più banale di questo mondo:

attraverso anche una Commissione della quale sono Presidente e della quale fanno parte tanti colleghi di maggioranza e opposizione, senatori e deputati, si è arrivati indubbiamente a svolgere un servizio positivo, anche in maniera *bipartisan*. Voglio ricordare che questa norma è contenuta nell'articolo 14 della legge di semplificazione n. 246 del 2005, che è stato posto in attuazione nel 2006 dal Governo Prodi

conclusione con l'attuale Governo. L'ampliamento dei termini, tra l'altro, è tale che mette nelle mani del Governo a partire dal 2014, quindi dopo la scadenza naturale di questa legislatura, la possibilità di intervenire. Perché questo emendamento è posto in questo articolo? In realtà, come relatore dei testi stralciati lo avevo previsto in altra sede,

con un riordino, se non di tutte, di buona parte delle materie oggetto di questa procedura di ricognizione, e poi di abrogazione, di norme già abrogate di per sé. Quindi, non aggiungiamo né togliamo nulla all'ordinamento. È stato inserito qui perché questa appunto con un riordino, quindi con la codificazione, che fino ad oggi ha prodotto già risultati importanti: ha ricordato prima il presidente Vizzini il codice dell'ordinamento militare, che rappresenta

in corso di perfezionamento anche il codice dell'agricoltura. Quindi, è indubbiamente una procedura sulla quale si è trovato, là di alcune scelte di merito, un consenso ampio, e si è ritenuto di potenziare, quantomeno nei termini, la delega. Quindi, non si tratta di cancellare il codice civile o il codice penale,

Se si vuole polemizzare su questo punto e in questa sede, io non ho alcuna difficoltà a far riprendere all'emendamento il posto che aveva, cioè all'articolo 19 invece che del tutto conforme allo spirito dell'articolo 43, che riguarda la codificazione, intervenire anche su questa procedura che - ripeto - ha trovato dall'inizio la condivisione però non abbiamo avuto occasione di ragionarvi in Commissione, mi rendo conto che un intervento, magari fatto per parti separate di un provvedimento molto complesso, possa generare quell'equivoco

perché i suoi rilievi non tolgono nulla all'eccezione che ho formulato. Infatti, l'eccezione di improponibilità attiene alla materia; l'ampiezza di intervento possibile da parte del Governo quale legislatore delegato nulla ha a che vedere con l'estraneità della materia. In ogni caso, non è vero che il Governo, quale legislatore delegato o titolare del potere di emanare regolamenti, potrà limitarsi solo a registrare l'intervenuta abrogazione di norme giuridiche. Ciò non è vero, perché il comma 14 citato dal collega Pastore prevede che l'intervento in sede di semplificazione normativa sia molto più esteso della semplice registrazione dell'intervenuta abrogazione, implicita

che ho menzionato è estranea all'oggetto e al titolo del provvedimento, non ha nulla a che fare con la materia dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Il codice civile regola - come è noto a tutti - il rapporto tra privati, e non tra la pubblica amministrazione

dall'oggetto del testo normativo in esame.

parere del Governo

Cerchiamo di ridurre il più possibile questo eccesso di delega in bianco, che consideriamo lesivo dell'autonomia delle

il Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud, in sintonia con il Governo e con il sottosegretario Augello, ritiene che con questo provvedimento si compia la scelta razionale di non voler inseguire con foga un generico progetto di semplificazione normativa della pubblica amministrazione, che porterebbe ad aumentare il numero di leggi e provvedimenti che compongono la «selva selvaggia» della semplificazione amministrativa e della sburocratizzazione che si è negli anni costituita. Sarebbe un ennesimo tampone non utile a niente, che porterebbe anzi la sicura conseguenza di aumentare la confusione e la poca chiarezza delle procedure a cui debbono attenersi i privati cittadini e, soprattutto, le imprese nel loro rapporto con lo Stato. Penso sia utile proporre una brevissima carrellata panoramica tra le leggi prese in considerazione da questo provvedimento, che da solo sottolinea, senza bisogno di grosse interpretazioni, la necessità di riformare la burocrazia e di adeguarla agli standard degli altri Paesi europei più avanzati.

Inoltre, di norma, la pubblica amministrazione agisce secondo le regole del diritto privato e questo è molto importante in uno Stato di diritto, quale il nostro. Il provvedimento riguarda inoltre le tempistiche che deve rispettare la pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi, l'istituzione della Conferenza dei Servizi e le norme che regolano l'accesso agli atti, all'insegna della massima trasparenza trasparenza possibile, in un'ottica non solo anticorruzione bensì anche di agevolazione del cittadino che ha necessità di ìnterfacciarsi con l'amministrazione statale e pubblica. Un altro importante provvedimento che viene preso in esame dall'articolo 43 riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che introduce l'importante novità della autocertificazione nella pubblica amministrazione. vi sono altri provvedimenti, tra cui i due decreti legislativi della cosiddetta riforma Brunetta che, in alcuni articoli, legiferano sulle norme che regolano il rapporto tra la pubblica amministrazione e gli utenti in materia di trasparenza, sia attraverso l'istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico sia imponendo l'accessibilità totale alle informazioni sul funzionamento di uffici e servizi della pubblica amministrazione per il pubblico. Questa accessibilità viene vista come forma di trasparenza nei rapporti tra il cittadino e l'amministrazione pubblica. Di fronte a tutti questi provvedimenti, più volte emendati e modificati, consci della necessità di uniformare ed aggiornare le norme che regolano i procedimenti amministrativi e la burocrazia in generale, soprattutto alla luce delle numerose e sempre innovative caratteristiche informatiche di cui la nostra società è sempre più dipendente, il Gruppo CN-Io Sud sostiene l'approvazione della delega al Governo per semplificare in maniera ordinata e radicale la pubblica amministrazione, riunendo ed aggiornando tutte le norme in appositi codici e testi unici. Inoltre, siamo sicuri che tutte le norme di semplificazione della burocrazia per le imprese costituiscono un importante volano per la ripresa economica che ancora stenta a perpetuarsi ed a riprendersi nel nostro Paese. È per questo quanto mai opportuno che dette norme non siano scollegate dagli altri provvedimenti in materia di sviluppo economico; considerato soprattutto che il decreto-legge n. 70, già approvato dalla Camera dei deputati, approderà a breve in Aula qui al Senato. Quindi, questi importanti provvedimenti che senz'altro recano carattere di urgenza in particolare per tutte le imprese operanti in territorio italiano,

su un provvedimento di 44 articoli. Alla fine di questo *iter* anche un po' macchinoso, lungo, come sono giustamente i lavori parlamentari - si discute in Commissione, si presentano emendamenti, ci si pensa sopra, si cambia idea, si cerca di far cambiare idea ai colleghi della parte avversa, ci si ingegna con i mezzi della persuasione e dell'interlocuzione dialettica,

e di questi 44 articoli se ne "stecchiscono" 43 e ce ne rimane uno solo, per votare. Che fine fanno gli articoli stralciati? Una parte vanno a finire in un decreto-legge, su cui probabilmente il Governo metterà la fiducia, in tal modo entrano in un universo chiuso in cui la possibilità di interlocuzione dell'Assemblea è praticamente ridotta a zero. Per altri articoli, che erano di relativa semplicità, si definisce un meccanismo barocco di costruzione di un'ulteriore delega al Governo, perché si ingegni a complicare la semplificazione. Su questa base, addirittura il titolo del provvedimento è doppiamente ironico: ironico perché la semplificazione è brutale (si passa da 44 articoli ad uno solo: più semplificazione di così si muore!); ironico perché dalla semplificazione si passa alla complicazione: si spostano gli articoli all'interno di un decreto-legge, si spostano altri articoli dentro una delega al Governo, e da qui nasce un'ulteriore complicazione. Semplificazione vera? No. In realtà è un procedimento a salti: due passi avanti e uno indietro, un passo avanti e due indietro, e alla fine si ha un risultato assai poco onorevole per un'Assemblea elettiva. Noi votiamo contro questa scelta, e la consideriamo esemplare, appunto, della rassegnazione dell'Aula nel consegnarsi ad una servitù volontaria verso il potere esecutivo.

Signora Presidente, colleghi senatori, un provvedimento intitolato originariamente alla semplificazione della pubblica amministrazione, portato avanti da una maggioranza che ne ha fatto - a mio avviso giustamente - un cavallo di battaglia, avrebbe dovuto vedere, nelle speranze mie personali, ma credo anche di tutto il mio Gruppo, una dichiarazione di voto assai più favorevole di quella che mi accingo a fare. In realtà, com'è stato ricordato, lo stralcio maxi, di 43 articoli su 44, depotenzia molto - per usare un eufemismo la portata di questo provvedimento. Il primo stralcio, il più rilevante, è motivato - a mio avviso, male - dall'introduzione di alcune norme semplificatrici nel "decreto sviluppo", e questo è stato

la semplificazione che si era inteso fare. Quindi, non solo è inutile, ma addirittura dannoso, anche nel momento in cui emargina il Parlamento, perché riconduce ad una successiva delega al Governo la possibilità di coordinare l'esito Il secondo stralcio è addirittura incomprensibile: articoli 41 e 42. La Carta dei doveri delle pubbliche amministrazioni è già discutibile che debba dar luogo ad un provvedimento separato rispetto a quello di cui oggi si parla e di cui si parla nell'articolo 43; è totalmente incomprensibile che la norma di delega debba essere diversa da quella della quale discutiamo e sulla quale votiamo oggi. Tuttavia, questi stralci sono stati votati, e noi di fatto ci troviamo a commentare esclusivamente l'articolo 43, al punto che il provvedimento nemmeno più si intitola alla semplificazione, ma alla codificazione delle norme sulla semplificazione, ed è un po' paradossale. Credo che la semplificazione richiami degli essenziali diritti di libertà dei cittadini e sia anche cruciale per la competitività delle imprese italiane che operano in Italia. La semplificazione è dunque un valore di libertà, ma è anche un valore economico, e come tutti i valori economici desume proprio il suo valore dalla scarsità. La semplificazione varrebbe molto in Italia, perché ce n'è poca, perché l'abbiamo

selvaggia di norme, ma come l'eliminazione di un fardello di regole e di norme inutili, ridondanti o addirittura dannose, che pure sono state introdotte da qualcuno (e, ahimè, sono state introdotte in prima istanza da decisori politici, e in seconda istanza da decisori burocratici che hanno desunto dai primi il loro potere, progressivamente crescente). Allora, la semplificazione in Italia dovrebbe avere qualcosa di Sun Tzu, fare un piccolo passo indietro per poi spiccare un grande balzo in avanti. Invece ha qualcosa di Kafka, nel senso che noi oggi introduciamo una norma che si limita a delegare qualcuno, che a sua volta delegherà qualcun altro - essenzialmente il Consiglio di Stato - per semplificare

Tuttavia, è uno dei necessari punti di partenza. La mia riflessione è un po' amara, ma non necessariamente polemica. Certo è che il Governo, che ha fatto - e ripeto giustamente - di questa una propria battaglia importante di principio, un vero e proprio cavallo di battaglia, a partire dalle elezioni e per tutto il prosieguo della legislatura, poteva davvero arrivare ad un risultato migliore. Si è parlato di un topolino partorito dalla montagna, ma temo che il topolino non riuscirà, come proverbialmente accade, a spaventare l'elefante, cioè la pubblica amministrazione. In questo senso, credo che l'Italia che lavora, l'Italia dei cittadini e delle imprese, l'Italia di destra come di sinistra, l'Italia dei lavoratori, degli imprenditori e dei pensionati, l'Italia che vive fuori di qui e che aveva un'altra idea di semplificazione non accetterebbe ciò che stiamo cercando di vendergli

*(LNP)*. Signora Presidente, spesso si parla con enfasi di cambiamento, esagerando la portata di episodi della politica e, al contrario, sottostimandone altri. Basti pensare che nei giorni successivi alla recente tornata di elezioni amministrative e all'indomani dell'esito referendario, la propaganda del centrosinistra ha dipinto alcuni risultati elettorali come fossero l'avvento di una primavera della società, provvidenzialmente giunta a risvegliare le coscienze dal plumbeo inverno berlusconiano. Così, guardando all'elezione di De Magistris a sindaco di Napoli, si è magnificato quel preteso vento di novità che, ahimè, oggi spira diffondendo il consueto olezzo dell'immondizia partenopea. Quanto alla capitale morale, la Milano liberata dalla retriva borghesia meneghina, cultrice di quegli *status symbol* offensivi della povertà terzomondiale, il primo atto pubblico del nuovo sindaco è stato precisamente il sopralluogo in uno dei più esclusivi e costosi *atelier* sartoriali di piazza San Babila. primo cittadino più amato dai *descamisados* dei centri sociali ha ordinato per sé alcuni abiti e camicie su misura, spendendo in pochi minuti quanto un lavoratore guadagna in parecchi mesi di fatica. *Nihil novi sub soli*, niente di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire con gli antichi se, al di là della demagogia, non si presentassero, di tanto in tanto, reali opportunità di cambiamento, segnali di svolta che attestino l'intenzione seria d'imboccare la strada attesa dal Paese. Ho ragione di ritenere che il provvedimento in esame, come tutti i precedenti e quelli che dovranno essere adottati, foriero di fatti e determinazioni, si inserisca nel filone di rinnovamento che attiene all'azione politica di questo Governo. Scorrendo il breve testo, finalizzato ad aprire la strada ai correttivi del malsano rapporto che nei decenni si è instaurato tra burocrazia e cittadini, verrebbe da chiedersi come mai tali misure, o analoghe, non siano state sin qui promosse da partiti di lunga consuetudine col Palazzo che, a parole, si proclamano democratici nonché paladini dei diritti dei cittadini e fustigatori delle prevaricazioni e, in questa circostanza, dimostrano per tali temi una premura mai concretizzatasi in precedenza. Eppure l'argomento è determinante. L'Italia, fatte le dovute eccezioni di luoghi e persone, porta il peso di una casta burocratica che gestisce il complesso di ostacoli imposti al Paese che lavora e produce. C'è da rimanere a bocca aperta nell'apprendere di certe inchieste giornalistiche da cui si evince come, in alcune Regioni, la diffusa disoccupazione giovanile sia, almeno parzialmente, dovuta al rifiuto delle opportunità lavorative che si presentano,

Sappiamo come l'attrattiva economica di tali posti non sia delle più appaganti, ed allora l'appetibilità di questa collocazione deriva da altri fattori psicologici che occorre rimuovere, tra questi l'assodata convinzione che all'addetto sia richiesta una scarsa sollecitudine nonché concessa una sorta di potere derivato, dato che il cittadino troppo spesso risulta in balìa degli innumerevoli lacci e lacciuoli amministrativi e di chi, in qualche misura e per il ruolo che gli compete, si arroga il potere di stringere o allentare quei cappi. Questioni ben presenti al legislatore, visto che nella logica e nell'ambito, molto esteso, della normativa in discussione ha trovato spazio la definizione di una Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche motivata, testualmente, dalla necessità di contrastare le molestie amministrative e assicurare l'effettività ai diritti delle imprese e dei cittadini. Si parla, dunque, di vessazioni da parte di soggetti remunerati dallo stesso contribuente che tali angherie subisce: una circostanza inaccettabile, scandalosa, indegna di un Paese civile. Situazione, peraltro, diffusa se la Commissione UE ha valutato in circa 70 miliardi di euro l'anno, pari al 4,6 per cento del nostro PIL, l'incidenza dei costi amministrativi causati dalla complicazione burocratica in questo Paese. Un autentico handicap, ritenuto tra le prime cause dello svantaggio competitivo italiano nell'ambito europeo e dell'area OCSE. Ad alcuni di questi impedimenti ora si guarda con misure *ad hoc*, premessa agli interventi che affronteranno il problema in maniera esaustiva, fornendo alla vita sociale e al mondo del lavoro quelle soluzioni che agevolano i rapporti con l'amministrazione. Dalla comunicazione unica per l'impresa, alla facilitazione per la cessione delle aziende, a certi automatismi negli appalti, sino alle misure sui trasporti eccezionali si coglie il *leit motiv* della semplificazione e dell'attenzione verso il cittadino che ritroviamo nelle direttive per gli per gli obblighi della pubblica amministrazione. Non possiamo, dunque, che accogliere positivamente questo provvedimento, così come abbiamo salutato quali cambiamenti di rotta quegli interventi del Ministro per la semplificazione normativa, che hanno messo ordine nella soffocante giungla legislativa, sfoltendola con decisione, consapevole della sentenza di Tacito, per il quale la corruzione dello Stato si riconosce dal gran numero di leggi. Così, in uno Stato a lungo afflitto da legislazione in gran parte pensata al fine di opprimere i cittadini, il vero cambiamento si ravvisa nella progressiva applicazione di norme concepite allo scopo di liberarli.

considerato anche il non affollamento di argomenti all'ordine del giorno. Il tema della semplificazione amministrativa, che conteneva talune soluzioni, alcune delle quali sicuramente migliorabili, è un tema importante che questa Camera avrebbe dovuto affrontare.

da processi decisionali inefficienti, dei quali si parla da molto, troppo tempo mentre la maggioranza, di tanto in tanto, si vanta parlando di sferzata all'economia, di competitività, di innovazione: tutte cose che tardano a venire. Il testo originario interveniva in molti comparti: in materia ambientale e paesaggistica (articolo 10), sugli infortuni sul lavoro, per i lavoratori dei settori del turismo e dello spettacolo, sul rilascio delle cartelle cliniche, per la trasparenza nella pubblica amministrazione, per le imprese. Insomma, tanti e tanti argomenti,

un provvedimento che richiederà l'espressione di un voto di fiducia da parte del Senato. Naturalmente, siamo assolutamente contrari a questo modo di procedere, al metodo che si è usato e al merito delle norme che potevano essere trattate. Nell'esercizio della delega, il Governo, che sarà tenuto ad assicurare il mero coordinamento formale delle disposizioni, evitando dunque qualsiasi tipo di intervento innovativo in proposito, aveva cercato di introdurre - pur comprendendo la buona fede e le motivazioni

nel più ampio complesso di una necessaria riforma della pubblica amministrazione, che non doveva comunque limitarsi a proclami e *slogan* (ma questo abbiamo visto fare in questi anni dai Ministri competenti, piuttosto che occuparsi dei singoli problemi per risolverli in un'ottica organica), questo procedimento dimostra certamente come si è mancata un'altra riforma, come la pubblica amministrazione che doveva essere oggetto di attenta analisi sia stata liquidata con provvedimenti di facciata, ovvero con provvedimenti che semplificano semplicemente riordinando il quadro normativo in modo, ahimè, confusionario e talvolta sovrapposto.

per optare, infine, per la strada della differenziazione, dell'analisi puntuale dei punti che andavano aggrediti per essere cambiati. E dunque tempo che lui stesso faccia un bilancio anche di questa sua impostazione che è stata pericolosa, inutile e perniciosa per una riforma della pubblica amministrazione. La prima strada sarebbe stata quella della trasparenza, che non si fa solo con le norme, ma anche con le tecnologie, con la reale possibilità di far accedere i cittadini agli atti amministrativi.

il testo che stiamo per approvare consta di un solo articolo, poiché gli altri articoli che formavano il testo originario seguono altre strade. Alcuni hanno hanno già trovato attuazione nel decreto-legge n. 70 del 2011, le cui norme sono già in vigore, sono state approvate con modificazioni dalla Camera e sono all'attenzione del Senato, che sta lavorando per l'approvazione definitiva

hanno in parte trovato attuazione ed in parte seguiranno un percorso proprio, dando luogo a un *iter* più snello che porti all'approvazione reale delle norme che andranno realmente a semplificare la pubblica amministrazione.

le norme che riguardano i principi generali delle amministrazioni pubbliche, un testo delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia di documentazione il decreto-legge n. 165 del 2001 (estremamente importante per il funzionamento della pubblica amministrazione, in particolare per quanto riguarda la dirigenza), il codice amministrativo digitale, più altre norme del decreto legislativo n. 150 del 2009, che si occupa in particolare dell'accesso alla pubblica amministrazione, ed altri ancora. Sarà così possibile per i per coloro che si trovano ad avere a che fare con la pubblica amministrazione avere, in un solo testo organico e coerente, tutte le norme che servono nei rapporti con la pubblica amministrazione. È questo un fatto estremamente importante, poiché i codici sono davvero un modo di semplificare i rapporti dei cittadini: sono un modo per porre le premesse anche per una riduzione del costo della pubblica amministrazione. Naturalmente queste norme dovranno trovare piena attuazione da parte della pubblica amministrazione stessa, a partire dai suoi dirigenti, che dovranno evitare di essere, a volte, coloro che fanno resistenza rispetto alla semplificazione che viene fatta per legge. In questo Parlamento, di leggi ci occupiamo, di leggi ci occupiamo, e il codice è sicuramente uno strumento di grande utilità. Un codice non viene fatto soltanto nel settore della pubblica amministrazione, esso si aggiunge ai numerosi codici che sono stati approvati negli ultimi anni: penso al codice dei contratti pubblici, al codice dei beni culturali, al codice del turismo, al codice dell'amministrazione digitale, al codice dell'ordinamento militare, al codice del consumo,

di un disegno di legge, bensì la sua portata. Questo testo è sicuramente positivo per i cittadini e per la pubblica amministrazione. Ritengo che facciamo bene il nostro lavoro portandolo a compimento, staccandolo dal resto del testo, che - comunque - in parte ha già avuto, e per il resto avrà, la sua approvazione nelle sedi proprie, secondo i rispettivi *iter* legislativi.

vera e propria succursale dell'ABI e dei banchieri, in particolare sulla vicenda definita Parentopoli, ossia l'assunzione per chiamata diretta, senza concorsi di pubblica evidenza, di amici degli amici, che ha generato assunzioni clientelari non dei migliori, ma dei peggiori dirigenti. Vede, signora Presidente, quando un commissario come Conti, ex dirigente bancario, persegue gli esclusivi interessi delle banche, eseguendo i *desiderata* dei banchieri (in particolare del signor Profumo), compie abusi sanzionati dai giudici di merito, come le corti d'appello, che poi sono suscettibili di azioni risarcitorie. Ma la prova più lampante di assunzione clientelare di parenti ed amici è rappresentata dalla Divisione legale CONSOB, composta dai signori Fabio Biagianti, Maria Letizia Ermetes e Paolo Palmisano. questi signori, adusi ad eseguire i *desiderata* e i condizionamenti interni, specie di alcuni banchieri che utilizzano il sistema delle porte girevoli tra la direzione generale dell'ABI e della CONSOB (Zadra e Sabatini), presentano ricorsi intrisi di così gravi errori da non superare neppure gli esami al primo anno di giurisprudenza. Vede, signora Presidente, risulta che siano stati assunti in CONSOB non pochi tra dirigenti e funzionari senza laurea e con selezioni pilotate da ragioni politico‑clientelari, senza tener conto delle disposizioni di legge.

che neanche abbiano effettivamente conseguito il diploma di laurea, e che non abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione forense. Mi avvio alla conclusione perché non riesco a capire su quali basi normative sia stato autorizzato l'avvocato Colavecchi, coadiutore della CONSOB, segretario della Commissione, a certificare la conformità delle copie vuote dei prefati documenti, quelli dei ricorsi in Cassazione, costellati di *omissis*, funzionali ad occultare le seriali malefatte. Vede, signora Presidente, la CONSOB è accusata di omessa vigilanza,

penale della procura della Repubblica di Parma. Chiedo, signora Presidente, che il Governo, e il Ministro dell'economia, che ha nominato Giuseppe Vegas presidente della CONSOB, venga in questa Aula e risponda a

distrutto un milione di famiglie e 50 miliardi di euro. Questa storia deve finire. Serve trasparenza e serietà.

di prendere in considerazione un argomento, che sottopongo all'Aula, assai delicato e certamente rilevante sotto il profilo delle forme istituzionali, ancorché siano depositati nelle sedi parlamentari diversi disegni di legge con firme diverse (cito solo i colleghi Butti, Perduca, con il quale ho persino concordato i temi di questo intervento,

materia che lo stesso Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua recente relazione annuale di qualche giorno fa, ha e cito, essere argomento meritevole di una consacrazione a livello di legislazione primaria con principi guida equilibrati.

metterebbe in atto una normativa, a mio modo di vedere, assai poco democratica, simile, per capirci, all'HADOPI francese ma che, detto in breve, istituirebbe una procedura senza giudice, secondo la quale si potrebbero sia erogare sanzioni, sia chiedere agli Internet *service provider* di rendere irraggiungibili i siti, ovvero di oscurarli. Solo in Cina e in Iran e parzialmente, in Francia, si arriverebbe a tanto, o si è arrivati a tanto. Il Parlamento si riappropri della sua funzione legislativa e si chieda al presidente dell'Autorità, Calabrò, di sospendere questa decisione in attesa di una iniziativa parlamentare.

Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta a una mia interrogazione, la 4-05235, presentata il 19 maggio scorso al ministro Sacconi. interrogazione riguarda i dipendenti del *call center* della società FESTA, del gruppo SNAI, leader noto a tutti nel settore dei giochi e delle scommesse, che ha sedi sia a Roma che a Lucca. In particolare, mi riferisco a quei lavoratori che si sono opposti alla proposta di rinunciare al contratto nazionale delle telecomunicazioni e di accettare invece un contratto aziendale, chiaramente con minori tutele. Il tribunale di Roma ha condannato la società FESTA per condotta antisindacale per aver firmato l'accordo con il solo sindacato Fistel-CISL, decretando le coesistenza di due tipologie contrattuali all'interno della stessa azienda. A pochi giorni da questa sentenza apprendiamo - ne ho qui la copia - che i lavoratori che non hanno sottoscritto l'accordo aziendale hanno ricevuto una lettera di licenziamento. Quindi, è un fatto davvero grave: l'atteggiamento di questa società è davvero deprecabile, e direi immorale. Sollecito pertanto il ministro Sacconi a intervenire immediatamente su tale situazione, che è davvero grave, e direi

a firma di 16 senatori, quasi tutti colleghi del Lazio, che riguarda due strutture di ricerca e cura a carattere scientifico che operano nella nostra città e nella nostra Regione: la Fondazione Santa Lucia e l'Istituto San Raffaele. Avevo chiesto che il Ministro venisse in Aula, a fronte di una situazione che diventa sempre più di emergenza, e non devo dirlo a lei, signora Presidente, che è attenta. Qualche giorno fa, l'autorità di pubblica sicurezza, nell'adempimento dei propri doveri, ha incriminato 22 medici di una di queste strutture perché hanno partecipato a una serie di manifestazioni. Sono giorni ormai che tra via Cristoforo Colombo e via Ardeatina ci sono manifestazioni di protesta. Da una parte, c'è il tentativo della Regione di venire incontro a queste esigenze; dall'altra, siccome sono tutti e due istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, c'è anche una responsabilità governativa. Avevamo chiesto al Ministro di venire a illustrare questa situazione, ma anche il richiamo fatto dalla Presidenza del Senato non ha raccolto nessuna

che devono trovare collocazione in altre strutture, e ad oggi la ASL competente territorialmente, la Roma H, non ha ancora provveduto ad alcuna iniziativa di tal genere.

Ho chiesto di sapere quali sono le iniziative che il Governo sta prendendo, e da parte del ministro Fazio c'è stato il silenzio. Voglio ricordare al ministro Fazio che non esiste solo la Lombardia, come Regione, ma anche la Regione Lazio.

un episodio invero minore rispetto a tanti altri più gravi nei rapporti tra Governo e Parlamento, ma che volevo segnalare perché è indice

trasporti Matteoli ha ritenuto di rispondere con una fotocopia della prima risposta. Può anche essere che la seconda interrogazione non sollevasse nel merito del giudizio che - come sempre - è opinabile. Dal punto di vista della forma,

alle signore che lavorano negli uffici con le imprese di pulizia. Non penso sia un grandissimo problema se nel calendario dei lavori del prossimo anno si terrà conto delle giornate lavorative, magari estendendo